Signor Presidente, come da lei anticipato, l'interpellanza riguarda la sorte della riforma Moratti sulla

- mi dispiace che questo non sia toccato in sorte anche al rappresentante del Governo che dovrà qui rispondere - abbiamo presente il dibattito che si è svolto in quest'Aula fino a qualche ora fa in tema di giustizia.

i due diversi schieramenti che si contrappongono in quest'Assemblea. Nella giornata di ieri, e in quella di oggi, abbiamo assistito non soltanto ad una contrapposizione civile, ma anche al tentativo di trovare dei punti d'intesa e di accordo che hanno portato alla sospensione di una seduta

è stata dunque una rappresentazione sofferta di due linee antitetiche, una delle quali è rappresentata dalla riforma approvata nella scorsa legislatura e l'altra, invece, dalla volontà di sospenderne gli effetti. A noi sarebbe piaciuto che la stessa rappresentazione fosse andata in scena per quel che concerne la scuola. caso ci troviamo di fronte ad una tematica che divide profondamente gli schieramenti. Nessuno nega la legittimità di questa differenza di

non possiamo negarlo certamente noi che, nella scorsa legislatura, abbiamo operato una riforma per cambiare quanto il precedente Governo, e in particolare il ministro Berlinguer, aveva fissato.

al servizio degli individui e chi invece ritiene che la scuola si debba riferire piuttosto alle comunità, in particolare alla comunità nazionale.

possibilità che diverse ipotesi pedagogiche ed educative entrino in concorrenza tra di loro. Deriva anche una diversità di fondo sul ruolo che lo Stato deve occupare per quel che concerne la scuola perché che lo Stato debba avere un ruolo importante nell'educazione nessuno lo metta in dubbio.

tutto ciò definisce un problema epocale. Io ritengo che, al cospetto dei cambiamenti sociali che interessano la nostra società che sempre più viene attraversata dalla presenza di

potessero confrontarsi, ricercare possibili punti di accordo e, nel caso, accertare una irriducibile diversità

(in particolare quelle che facevano riferimento a quella visione personalistica, che ritengo sia al fondo di una delle due visioni competitive che per ragioni di brevità ho dovuto schematizzare) siano state

il contratto collettivo è fonte secondaria di produzione di norme e, in mancanza di un atto di indirizzo del Governo, ai sensi della legge n. 165 del 2001, esso non ha la possibilità di abrogare una norma di grado primario, come invece è avvenuto.

assume un insopportabile sapore di sopruso laddove si pensi che la contrattazione collettiva prevista dalla cosiddetta che si sarebbe dovuta svolgere in sede ARAN, è stata bloccata dai sindacati nel corso di tutta la scorsa legislatura, sebbene più volte sollecitata. Dunque,

l'auspicato avvento di un Governo amico (che, tra le altre cose, negli ultimi mesi della legislatura appariva più probabile di quanto poi le urne hanno rappresentato)

della normativa che non era considerata con occhio favorevole dai sindacati. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo,

Si chiede, pertanto, se il Governo ritiene veramente che con una contrattazione collettiva si possano abrogare

in un metodo, quello della democrazia competitiva e conflittuale, o se piuttosto ritenete indulgere verso un'altra concezione

e magari lo scontro, tra le posizioni legittimamente sostenute dal Governo e quelle che possono invece maturare all'interno delle Aule del Parlamento.

rammento che l'accordo in sede ARAN è stato sottoscritto il 17 luglio da tutte le organizzazioni sindacali rappresentative, dalla GILDA allo SNALS, alle organizzazioni confederali, che hanno espresso in merito consenso unanime. Si tratta di una sequenza contrattuale sottoscritta ai sensi dell'articolo 43 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, siglato il 24 luglio 2003. Resto nel merito dello strumento giuridico, perché lei, senatore Quagliariello, mi ha particolarmente sollecitata questo punto. Voglio ricordare che questo strumento, previsto dal contratto, prevede che la disciplina contrattuale sia suscettibile delle modifiche che in via pattizia si renderanno necessarie in relazione all'entrata in vigore della legge n. 53 del 2003 e delle connesse disposizioni attuative.

che incide profondamente sull'organizzazione del lavoro del personale della scuola, senza aver stipulato preventivamente con i sindacati un accordo sui contenuti delle modifiche dell'organizzazione del lavoro; ciò era tanto chiaro che si riconosceva espressamente tale necessità. La fonte giuridica del ruolo della sequenza contrattuale si trova all'articolo 1, combinato con l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale stabilisce testualmente che: "Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche o categorie di essi possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario".

Inoltre, qualora una legge decida che le sue norme o le norme di riferimento non possano essere derogate, deve espressamente indicare l'inderogabilità. Questa condizione non si riscontra nella legge n. 53 e quindi è confermato il principio di derogabilità, che costituisce, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001, "principio fondamentale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione". Tutto ciò per sottolineare l'auspicio del Governo affinché vi siano accordi e concertazioni di carattere preventivo e che solo in via straordinaria siano utilizzati questi strumenti

Nel merito, vediamo poi su quali norme si attesta la sequenza contrattuale, ovviamente norme rigorosamente attinenti alla organizzazione del lavoro:

Ovviamente la norma sul *tutor*, una funzione che viene attribuita ad uno dei docenti del gruppo classe, è collocata pienamente all'interno della disciplina relativa all'organizzazione dell'attività educativa e didattica e all'assegnazione dei docenti nelle classi. Quindi, è posta all'interno delle disposizioni del Testo unico in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994.

La scelta adottata dall'accordo ARAN è finalizzata a conferire una più razionale organizzazione della funzione tutoriale. Infatti, i compiti connessi alla figura del *tutor* vengono spalmati su tutti i docenti, facendone una funzione che fa capo a ciascuno di essi nell'ambito dei vigenti istituti ed obblighi contrattuali. Pertanto, già dall'anno scolastico 2006‑2007 nulla viene innovato o modificato rispetto a quanto già previsto dagli articoli 24 (funzione docente), 25 (profilo professionale) e 26 (attività di insegnamento) del vigente contratto collettivo di lavoro. In sostanza, noi riportiamo quella funzione nell'alveo individuato dalle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro. Tale scelta evita che si debba individuare un docente con maggior carico orario nei primi tre anni delle scuole primarie, in violazione del principio di pari responsabilità di tutti i componenti del *team* didattico. Numerose pregresse esperienze legislative e contrattuali hanno in realtà dimostrato che qualunque processo di innovazione imposto dall'alto, senza un processo di condivisione da parte dei docenti, produce nelle scuole resistenze o adempimenti puramente burocratici e formali che non migliorano affatto la qualità del processo di insegnamento ed apprendimento, riducendosi spesso a risposte meramente cartacee. Vogliamo invece puntare, anche attraverso la sensibilizzazione e la formazione dei docenti e la collaborazione delle associazioni dei genitori, a ricostituire un clima di responsabilizzazione condivisa rispetto alle funzioni dell'orientamento, dell'assistenza all'alunno, del rapporto con i genitori, della documentazione dei percorsi didattici, funzioni che devono necessariamente coinvolgere indistintamente tutti i docenti, ciascuno per la propria disciplina e come componente del *team* educativo. Diverso è ovviamente il discorso sull'opportunità di promuovere funzioni di coordinamento e di organizzazione del lavoro che le scuole sono invitate ad incentivare, naturalmente nell'ambito dell'autonomia scolastica

del precariato. Questo è l'obiettivo che vogliamo perseguire. Preliminarmente va precisato che tali contratti sono previsti dal regolamento sull'autonomia approvato con decreto legislativo n. 275 del 1999 e si riferiscono ad insegnamenti aggiuntivi, espressione di qualificate professionalità esterne. Questi contratti sono in realtà già vigenti nel nostro ordinamento, secondo la disciplina dell'articolo 40 del decreto ministeriale n. che è il regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche, il quale affida la regolamentazione dell'istituto giuridico all'autonomia degli organi delle singole istituzioni scolastiche nell'ambito delle risorse finanziarie di cui le stesse dispongono. I contratti di prestazione d'opera trovano, del resto, da tempo attuazione soprattutto negli istituti di istruzione secondaria superiore. L'istituto giuridico, nella parte abrogata, costituiva in realtà un ibrido giuridico in base al quale venivano imputate a risorse finanziarie delle scuole, peraltro di norma insufficienti per pagare questo tipo di prestazioni, prestazioni didattiche obbligatorie per gli alunni che esercitano l'opzione, costituenti cioè a tutti gli effetti ore curricolari. Ricordiamoci che le ore opzionali erano obbligatorie e quindi costituivano parte del *curriculum*, e questa è l'anomalia che era stata evidenziata anche in sede di relazioni sindacali. L'applicazione del medesimo istituto giuridico avrebbe in concreto determinato una forte conflittualità, in quanto veniva a mascherare in realtà un rapporto di lavoro dipendente, organicamente inserito, anche ai fini delle valutazioni, nel curricolo obbligatorio degli alunni. Pertanto, l'applicazione di detto istituto avrebbe determinato una surrettizia forma di ulteriore nuovo precariato, che il Governo è invece intenzionato a ridurre e progressivamente ad eliminare. E tutto ciò senza aver concordato criteri trasparenti per la scelta dei docenti e in mancanza della preventiva definizione dei titoli per lo svolgimento di tali attività didattiche, che avrebbero dovuto essere definiti con decreto interministeriale. Infine, riguardo agli anticipi nella scuola dell'infanzia, l'accordo ha disapplicato tale istituto, in quanto allo stato non sussistono i presupposti richiesti dalla legge n. 53 del 2003. Manca, infatti, la definizione delle figure professionali necessarie (sono docenti, sono ATA, sono assistenti dell'infanzia del Comune?), la pur prevista specifica disciplina degli organici (meno alunni nelle classi con gli anticipatari) e, soprattutto, il quadro degli accordi con la Conferenza Stato-Regioni per assicurare tutte le condizioni a regime per la disciplina contrattuale a livello nazionale di eventuali figure professionali statali. Resta intesa ovviamente, per quel che riguarda l'anticipo, la possibilità di accordi locali per sperimentazioni da effettuare in presenza di tutte le condizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 59 del 2004,

la sequenza contrattuale punta a ristabilire un clima, io dico, di serenità nelle scuole e di confronto con le organizzazioni sindacali; oserei dire che può anche portare ad un clima di maggiore serenità dal punto di vista della legalità delle azioni che vengono svolte all'interno delle scuole. Credo che i processi di mutamento veri, che incidono sulla qualità della scuola e sul futuro della stessa, debbano assolutamente partire sempre dal basso, con un'ampia condivisione da parte degli operatori della scuola, che su queste norme non c'era stata, e soprattutto con un vero processo di concertazione con le parti sociali, le organizzazioni sindacali, la Conferenza Stato-Regioni, le autonomie locali, perché è solo da questi processi che riusciremo ad operare (mi auguro con un ampio dibattito nel Senato e nelle Aule parlamentari) un vero processo di cambiamento del nostro sistema scolastico.

soddisfatto della risposta del Governo perché chi leggerà gli atti parlamentari - quei pochi cultori della materia - comprenderà dalle parole del vice ministro Bastico che in realtà tutte le preoccupazioni presenti nell'interpellanza erano fondate. anzitutto che, per quel che concerne i rapporti tra il Legislativo e l'Esecutivo, il fatto che ci fosse l'unanimità delle organizzazioni e delle sigle sindacali in sede ARAN non motiva alcunché. Credo che su questo sarà d'accordo anche lei; se una decisione veniva assunta all'unanimità in sede di Camera dei fasci e delle corporazioni, non per questo era una decisione assunta attraverso un metodo di democrazia In secondo luogo, per quel che concerne la legittimità degli atti, ritengo che l'interpretazione che lei ha dato, sia della normativa primaria, sia del legge n. 165 del 2001, è un'interpretazione, diciamo così, estensiva, forse un po' troppo generosa: perché né il termine «modifica», né tanto meno quello della «deroga»,

andate ben al di là delle considerazioni di carattere legislativo. Hanno investito una filosofia complessiva della riforma del sistema scolastico assolutamente legittima, ma che proprio per la sua rilevanza e per la sua legittimità avrebbe dovuto risuonare innanzitutto all' interno delle Aule parlamentari.

l'invito finale da lei rivolto affinché quelle argomentazioni possano trovare spazio nelle discussioni del Parlamento

dal nostro Regolamento - presentare questa interpellanza con procedura abbreviata per fare finalmente chiarezza su una questione, su un fatto, su un problema che sta sostanzialmente dilaniando, lacerando e spaccando trasversalmente la città di Brindisi e l'intera provincia. Mi riferisco alla questione del rigassificatore. La storia della realizzazione di questa infrastruttura credo sia sufficientemente nota.

Tale decreto deriva, nasce e assume la propria legittimazione sulla scorta di un parere positivo espresso - ovviamente in data precedente rispetto al decreto medesimo dalla Conferenza dei servizi, nel corso della quale ebbero ad esprimersi positivamente, tra gli altri, la Regione Puglia, la Provincia e il Comune di Brindisi. il mutamento della guida politica di questi tre enti, sostanzialmente è venuta a cambiare anche la posizione a proposito della realizzazione del rigassificatore.

abbiamo cercato di assumere una posizione diversa rispetto alle due: abbiamo cioè detto in maniera molto chiara che eravamo favorevoli ai rigassificatori, perché c'è un problema energetico con il quale dobbiamo fare i conti;

ideologica - si potesse individuare un progetto alternativo di sviluppo per la città. Sull'argomento, che pure ci affascinava, chiedemmo - come chiediamo tuttora - quale fosse sostanzialmente questo nuovo modello di sviluppo e in quanto tempo si realizzasse, visto che Brindisi si trova a vivere una stagione pesantissima sotto il profilo sociale, dello sviluppo e occupazionale. In tutto questo periodo, mentre il di Alleanza Nazionale ed io personalmente invocavamo il dialogo istituzionale, cercando di evitare una rottura tra le istituzioni locali e le istituzioni nazionali, il Governo, questo Governo, non ha assolutamente fatto la sua parte. a differenza del Governo di centro‑destra, che aveva assunto sulla questione una posizione condivisibile o meno, ma sicuramente chiara, con il sì al rigassificatore, questo Governo si è invece caratterizzato fino ad oggi per l'ambiguità delle posizioni espresse non dai singoli parlamentari, ma dagli stessi esponenti dell'Esecutivo. E' di ieri la posizione espressa dal ministro dell'ambiente Pecoraro Scanio, che ha dichiarato da Bari che se il Governo sta ancora lavorando ad un'eventuale modifica del decreto di autorizzazione sulla realizzazione del gassificatore, ciò avviene grazie al Ministero dell'ambiente perché altrimenti il Governo avrebbe già detto che era tutto a posto. Ebbene, di fronte alla posizione ben definita di Pecoraro Scanio c'è

rigassificatore. A questa situazione di grande confusione aggiungiamo che pochi giorni fa si è tenuto qui a Roma un incontro tra le istituzioni locali ed esponenti del Governo nazionale proprio per definire, sia sotto il profilo tecnico

intellettuale, in cui versa questo Governo sulla materia. Intanto, sotto il profilo nazionale, continua ad sussistere, in maniera veramente forte e virulenta, il problema della capacità energetica del nostro Paese, sotto il profilo strettamente locale, la città continua a dividersi ancora di più ed esponenti politici di non secondario piano hanno già detto in maniera molto chiara che, qualora le cose non dovessero andare secondo i loro intendimenti, scenderanno in piazza. che ci troviamo di fronte ad una situazione pericolosissima, anche sotto il profilo dell'ordine pubblico; significa che non è consentito a nessuno - e quindi neanche a questo Governo - di poter ritenere di perdere ancora tempo nelle decisioni.

e chiedo al Governo di conoscere quale sia la posizione su questa materia controversa e più specificamente se il Governo medesimo intenda confermare o meno il decreto n. 17032 del 21 gennaio 2003 con il quale fu autorizzata la costruzione e l'esercizio di un rigassificatore a Brindisi in località Capo Bianco. Che cosa mi attendo dal Governo oggi? Mi attendo un atto di onestà politica, una manifestazione di senso di responsabilità e anche una prova di coraggio, perché non vorrei che in quest'Aula accadesse ciò che è accaduto ieri nell'altro ramo del Parlamento, quando, in maniera molto pavida, il Governo non si è assunto la responsabilità di decidere e di indicare una via precisa sulla materia. Questa mattina, leggendo la rassegna stampa, ho letto ed apprezzato molto un articolo di un nostro collega, il senatore Andrea Manzella, un articolo bellissimo il cui titolo era «Il Parlamento muore». Ecco, io dico subito al Governo che il Parlamento muore nel momento in cui si fugge dalle responsabilità, nel momento in cui non si decide, nel momento in cui in cui si snatura il ruolo di questa Camera.

e non preso in giro come è accaduto ieri nell'altro suo ramo, presso la Camera dei deputati, che possa essere rispettato nella sua funzione, ma più che il Parlamento, più che quest'Aula e più che lo stesso parlamentare, siano rispettate le popolazioni brindisine, che da questo Governo vogliono una risposta chiara su un argomento di straordinaria rilevanza per il loro futuro. Signor Presidente, voglio ringraziare il senatore Curto per le preoccupazioni che ha espresso voglio anche dirgli che siamo piuttosto dispiaciuti per la non tempestività della risposta, perché le questioni che sono poste all'attenzione del Governo e del Parlamento attraverso la sua interpellanza, sono questioni molto serie, che riguardano il futuro di una città importante della Puglia, riguardano la sicurezza energetica del nostro Paese, riguardano anche la certezza che va data ai cittadini e alle istituzioni circa il metodo che negli atti è necessario consacrare continuamente per quanto riguarda la tutela della salute e la tutela dell'ambiente. Il senatore Curto nell'interpellanza ha riassunto in maniera analitica, precisa e puntuale l'intera vicenda e nell'illustrazione ha rappresentato i motivi di turbamento, di smarrimento, di divisione che oggi sono riscontrabili nella città di Brindisi e ha segnalato come quegli enti locali che in sede di Conferenza di servizi avevano espresso il proprio assenso alla realizzazione di un'opera importante qual è il rigassificatore, successivamente, anche per effetto delle mutate maggioranze che si sono determinate, hanno cambiato opinione. Ma mi chiedo e chiedo al senatore Curto: la mutazione di posizione è figlia di un pregiudizio politico, o raccoglie una preoccupazione che la città esprime in ordine al proprio futuro, che deve guardare sì allo sviluppo, deve guardare sì all'accrescimento delle opportunità di natura industriale e di occupazione, ma che deve poter fare tutto questo tutelando l'ambiente e preservando la salute dei cittadini? L'amministrazione comunale di Brindisi, l'amministrazione provinciale e, da ultimo, la Regione Puglia, con un voto espresso all'unanimità hanno posto un problema di coerenza del procedimento autorizzativo con il quadro normativo fissato a livello comunitario. Non c'è dubbio che il rigassificatore non è ricompreso tra le opere per le quali è prevista espressamente la procedura di valutazione d'impatto ambientale e tuttavia le opere complementari e connesse al rigassificatore, trattandosi di opere impattanti, devono essere sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, la quale valutazione può esprimersi in forma abbreviata, accelerata o in forma analitica, compiuta attraverso un dibattimento pubblico, che è la parte rilevante che la direttiva comunitaria ha voluto fissare definendo la procedura di valutazione d'impatto ambientale. Ebbene, in questa fattispecie il Ministero dell'ambiente ha ritenuto soddisfacente la procedura abbreviata, caratterizzata dalla fase di *screening*, senza procedere alla valutazione di impatto ambientale che avrebbe comportato il pubblico dibattimento, la possibilità, cioè, di mettere a confronto le preoccupazioni e le richieste di cautela di attenzione che i portatori di interessi collettivi avrebbero potuto rappresentare. Ebbene, i ricorsi e le posizioni degli enti locali fondano su questi presupposti. Riteniamo che tali preoccupazioni siano legittime e che i dubbi e le perplessità vadano fugati. convinti, infatti, che anche le scelte che appaiono più complicate e difficili risultano sopportabili solo in ragione di un procedimento rigoroso, improntato, cioè, al rispetto puntuale, analitico delle norme comunitarie ed ispirato al principio di precauzione. Su questa vicenda sono in corso azioni e pronunciamenti che devono essere determinati da parte degli organi della Comunità europea, interessati per un presunto atto di violazione delle norme stesse. Ha ragione il senatore Curto: la città ha bisogno di certezze e il Governo non vuole rifuggire dalle proprie responsabilità.

per garantire il bilancio energetico del nostro Paese e per liberarci da una forma di dipendenza nell'approvvigionamento delle fonti primarie. tuttavia, che tutto ciò debba essere realizzato nel rigoroso rispetto delle norme, applicando le procedure più rigorose per tutelare la salute e l'ambiente. In questo senso, quindi, non possiamo che esprimere un pronunciamento preciso in ordine al fatto che gli atti emanati in coerenza con il quadro normativo ordinamentale siano efficaci fino ad atti che ne possano inficiare l'efficacia.

e che quel problema non appartiene al conflitto politico o elettorale, che pure si genera e che è legittimo e va compreso nelle nostre realtà, essendo le amministrazioni interessate di diverso orientamento politico ed essendo stato espresso all'unanimità il voto da parte del Consiglio regionale della Puglia. Segnaliamo un atteggiamento di prudenza, com'è stato fatto ieri alla Camera, in relazione alla necessaria attività di verifica, che deve essere effettuata - esattamente come il ministro Pecoraro Scanio ha annunciato - da parte degli organi che hanno la responsabilità e la titolarità nella tutela ambientale. Per questo motivo, considerato che l'impianto è autorizzato e che sono in corso i lavori, non abbiamo alcuna difficoltà nel dire che l'unica possibilità che la disciplina comunitaria offre è quella costituita dal giudizio di compatibilità emesso in corso di realizzazione dell'opera, la cosiddetta VIA postuma, se vogliamo dare certezza ai cittadini e alle istituzioni locali. La valutazione di questa possibilità è rimessa esclusivamente all'autorità competente a valutare gli effetti ambientali dell'opera che sola può, riesaminando l'interesse pubblico di salvaguardia ambientale, su tale base, chiedere la revoca del provvedimento e non il suo annullamento, essendosi perfezionato il procedimento che si è concluso con l'autorizzazione; revoca che potrebbe essere giustificata solo in presenza di sopravvenute diverse conclusioni, scaturenti dalla valutazione di impatto dell'opera sull'area territoriale di Brindisi. Alla luce di queste considerazioni, vanno interpretate e spiegate, in un quadro di assoluta coerenza, le posizioni espresse dal Ministro dell'ambiente che ha la titolarità in ordine ai procedimenti di tutela ambientale e quanto riferito nella giornata di ieri presso la Camera dei deputati.

che il soggetto titolato a rilasciare l'autorizzazione è stato il Ministero delle attività produttive, trovo difficoltà a comprendere come quel provvedimento possa essere revocato da un Ministero diverso, da un organo di Governo diverso. Sono molto sbalordito anche perché, di fatto, lei ha rivolto a me personalmente alcune domande, alle quali posso rispondere con grande franchezza: siamo tutti preoccupati, non solamente a Brindisi, ma nel nostro Paese della situazione ambientale e siamo tutti impegnati a fare in modo che sviluppo e tutela dell'ambiente coincidano, senza lasciare spazi a chi vuol fare sviluppo disinteressandosi dell'ambiente, ma anche non lasciando assolutamente spazio a chi dell'ambiente ne vuol fare solamente una battaglia ideologica per fermare lo sviluppo. Di fatto, credo che bisogna creare le condizioni per fare ragionamenti veramente seri,

non mi sarei mai aspettato una critica rivolta al Ministero dell'ambiente della passata legislatura, quantomeno per un motivo: non solamente perché sono convinto della legittimità

ma anche perché quella legittimità è stata in più occasioni espressa da vostri autorevolissimi esponenti, compreso il ministro Bersani. In più circostanze, egli ha infatti sostenuto che le procedure che portarono al rilascio di quell'autorizzazione sono perfette, perfette, efficaci e, soprattutto, corrette sotto il profilo procedurale e di merito. Queste sono le ragioni per cui, di fronte a situazioni di questo genere, ribadisco che incalzerò il Governo,

perché rispettiamo il Sottosegretario e i Ministri più o meno competenti in questa materia, ma ci costringerete a chiedere qui la presenza del Presidente del Consiglio perché non è più possibile, non è più tollerabile, non è più ammissibile che su un argomento di così straordinaria rilevanza le voci all'interno di un Esecutivo possano essere più di una e tutte discordanti. È grave il danno che state arrecando al Paese; è gravissimo il danno che state arrecando alla collettività.

e, in relazione a questi, alle più generali intenzioni dell'Esecutivo in merito alle politiche di governo dei flussi migratori e di riforma della connessa disciplina relativa al riconoscimento dei diritti di cittadinanza. Innanzitutto, è bene ricordare che la situazione di via Anelli a Padova purtroppo non è unica: altre *enclave* urbane hanno registrato una situazione di diffusa criminalità

nelle dinamiche politiche di quella città, tanto da partecipare apertamente alle primarie che hanno condotto all'individuazione del candidato dell'Ulivo.

Devo far riferimento a queste componenti della stessa coalizione che governa Padova e che sono state protagoniste di questi intollerabili scontri in città, perché la presenza di componenti radicali di tale natura può spiegare la ragione per cui l'amministrazione comunale di Padova è apparsa incerta rispetto ad un accordo di programma realizzato dall'amministrazione precedente, guidata dalla signora, oggi parlamentare, Giustina Destro.

tanto da condurre allo smantellamento delle stesse palazzine che - come precisato - costituiscono un ambito nel quale la legge dello Stato si è rivelata inefficace e che avrebbe dovuto condurre, attraverso l'intervento dell'ATER e della Regione, alla ricollocazione dei cittadini colà residenti, ma in condizioni di regolarità, all'individuazione degli irregolari con i conseguenti provvedimenti di espulsione e alla ricostruzione di un tessuto urbano qualificato e soggetto al controllo dello Stato. A questo programma non è stata data immediata esecuzione, tanto che si è arrivati all'edificazione del muro come disperato tampone

la certificazione di un'impotenza dell'amministrazione locale, la certificazione di una situazione di straordinario disagio per le persone per bene che abitano in quel territorio e che hanno il diritto di vivere nelle condizioni nelle condizioni proprie di una società civile. Vorrei ricordare che alla vicinissima Treviso, città dalla quale provengo, la Caritas ha recentemente riconosciuto - e mi permetto di considerarla a questo riguardo fonte non sospetta - il primato del processo di integrazione sotto i vari profili in

i flussi migratori hanno trovato, ove più ove meno, ma complessivamente, ragioni di integrazione; è una situazione che può e deve essere rimossa. Qual è l'intenzione del Governo a questo proposito e quale il giudizio del Governo nei confronti dei movimenti della sinistra antagonista che aggiungono problema a problema? Quale l'intenzione dell'Esecutivo in riferimento all'accordo di programma tra Comune, Regione e Governo? Quale la disponibilità ad investire risorse, posto che quelle a suo tempo ipotizzate possono probabilmente essere venute meno proprio per i colpevoli ritardi che si sono prodotti a tale riguardo, determinati, come ho detto, da incertezze connesse alle caratteristiche della coalizione che governa Padova?

ha parlato di una volontà di riforma quanto al governo dei flussi migratori. Sappiamo che, per quest'anno, si è adottata colpevolmente la decisione di una sanatoria di fatto, perché l'allargamento della quota al totale delle domande presentate ha il significato di una sanatoria a piè di lista. Ciò ha costituito, a nostro avviso, un segnale di attrazione per flussi clandestini che, non a caso, si sono prodotti in misura ben più consistente rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ci sembra colpevole che si voglia, da un lato, dare un segnale di permanente sanatoria a piè di lista e quindi di riproduzione di flussi migratori subiti e, dall'altro, collegare a tali flussi diritti di cittadinanza

attua fino in fondo quella legge Bossi-Fini che si vuole cambiare nonostante il 2006 sia il primo anno di compiuta implementazione della stessa. Mi riferisco soprattutto allo strumento principe individuato e cioè il regolamento di attuazione della legge che consiste nella formazione e selezione dei lavoratori nei Paesi di origine. Tale selezione viene realizzata a cura delle associazioni che rappresentano i datori di lavoro o, nel caso delle famiglie, da quelle riconosciute reti *non-profit*, soprattutto ecclesiastiche, per le famiglie costituiscono un punto di riferimento, in modo che si possa realizzare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro a distanza rispetto a persone che ancora sono nei Paesi di origine e che nei Paesi di origine hanno la possibilità di partecipare a corsi di formazione che danno luogo a possibilità di selezione, soprattutto se sostenuti da accordi tra il Paese ricevente, il nostro, e i Paesi che cedono flussi

con le intenzioni che porterebbero a ingressi senza la necessità di un contratto di lavoro e tantomeno di una casa o della conoscenza della lingua e in aggiunta la prospettiva di diritti di cittadinanza riconosciuti a flussi con queste caratteristiche dequalificate - per i quali cioè non vi è stata un'attenta verifica delle professionalità per un verso e delle provenienze geopolitiche per l'altro con i conseguenti problemi di possibile esclusione sociale

di rigorosa gestione dei flussi e di rigorosa conduzione dei processi di reale integrazione. Infatti, l'incontro tra il Paese d'accoglienza e i migranti è un percorso inesorabilmente aspro che deve essere condotto attraverso forme rigorose, le uniche che possono costituire il presupposto per una larga condivisione del riconoscimento di diritti di cittadinanza.

nel contenuto della sua illustrazione ho trovato un ampliamento del tema *decidendum* proposto dall'interpellanza e che comunque cercherò di seguirla

spiegare il senso, il tenore dell'interpellanza, che riguardava essenzialmente le politiche che si intendono seguire e realizzare rispetto al grande tema dell'immigrazione, a partire, come dicono i senatori che hanno firmato l'interpellanza, da alcuni episodi di cronaca che sono avvenuti a Padova nel mese di luglio scorso. A questo gli stessi senatori hanno aggiunto una richiesta ulteriore di conoscenza e di considerazione di considerazione delle linee d'intervento che il Governo intende porre in essere per il recupero della legalità e della coesione sociale di aree urbane degradate, anche a causa della criminalità, e hanno proposto alcuni quesiti che riguardano la più complessiva azione di governo delle politiche migratorie. Credo che proprio l'esperienza di Padova e, specificamente, del complesso di via Anelli, ci consenta di dire che le esperienze di emarginazione e di degrado che si realizzano o si possono realizzare nelle nostre città, esperienze che coinvolgono sempre di più le famiglie di immigrati, esperienze che raccontano vicende delittuose che rendono insicura la vita dei residenti, siano essi immigrati o italiani, richiedono una risposta che unisca gli interventi di prevenzione e di contrasto alla criminalità con azioni positive di recupero sociale ed urbano, anche per impedire che si creino dei luoghi di esclusione. La storia di via Anelli, infatti, è quella di un complesso residenziale composto da sei palazzine, per un totale di 286 piccoli appartamenti, che - come il senatore Sacconi sa - erano originariamente destinati agli studenti. Nel tempo, tuttavia, quel complesso ha subìto un progressivo degrado, anche a causa di un cambiamento della composizione sociale causato dalla tendenza dei proprietari a massimizzare la rendita degli immobili affittandoli a più persone fino a sovraffollarli. Ciòha condotto ad un grave deterioramento dello stato degli immobili, ad un decadimento graduale accompagnato da atti di inciviltà, danneggiamenti, vandalismi e anche da manifestazioni criminali ben più rilevanti, come quella cui fa cenno l'interpellanza. Ricordo che il complesso di via Anelli è arrivato ad ospitare circa 750 stranieri, in prevalenza di origine nigeriana e maghrebina. Tale situazione ha indotto l'attuale amministrazione comunale a programmare, già dal suo insediamento, specifici interventi per il recupero dell'area, che erano rimasti fin lì inattuati e che sono stati concretamente avviati a partire dal 2004. Il lavoro dell'amministrazione è stato affiancato dalla rigorosa e costante attività di controllo dell'area da parte delle forze dell'ordine, capaci di realizzare un reale coordinamento, una sinergia favorita dall'intesa positiva tra il prefetto e il questore. Sono state contate, solo negli ultimi dodici mesi, 22 operazioni straordinarie con 133 arresti. Lasera del 26 luglio, in particolare, l'immediato intervento delle forze dell'ordine ha scongiurato lo scontro tra gruppi contrapposti di origine maghrebina e nigeriana, in lotta, pare, per il controllo del mercato degli stupefacenti nella zona. L'operazione ha consentito l'arresto di 21 maghrebini, l'espulsione di 22 nigeriani, il sequestro di circa due chilogrammi di stupefacenti e di numerose armi da taglio. Sono stati identificati 172 stranieri e perquisite due palazzine. L'episodio ha, inoltre, indotto a rivisitare i dispositivi di prevenzione e controllo del territorio nella zona: a tal fine è stata disposta la chiusura al traffico

Per quanto di sua competenza, l'amministrazione comunale aveva già ridotto gli elementi di tensione nel complesso residenziale liberando in fasi successive, a partire dal febbraio 2005, tre delle sei palazzine e procedendo, quindi, alla nuova sistemazione degli inquilini in diverse zone della Città. Il progetto, che dovrà proseguire, come finora è avvenuto, attraverso la collaborazione con l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale, prevede un prossimo trasferimento di altre 40 famiglie fino al totale successivo sgombero di tutti gli appartamenti. La politica adottata dall'amministrazione comunale è riuscita finora a raccordare gli interventi di recupero dell'area

affidate dall'ente locale ad una cooperativa perché segua il loro inserimento dentro gli stabili di nuova abitazione anche con un'attività di mediazione culturale svolta per favorire la buona convivenza con i cittadini già residenti. Ma rispetto a tutto questo, ciò che ha maggiormente attratto l'attenzione dell'opinione pubblica, che ha suscitato dibattito con contestazioni e condivisioni (un'ampia condivisione e contestazioni anche accese) è stata certamente la decisione dell'amministrazione comunale di sostituire la vecchia e logora recinzione metallica con una recinzione con lastre in lamiera, quella che, con ampia eco mediatica, è stato definita «il muro di via Anelli». L'intervento è stato limitato al confine tra il complesso residenziale e via De Besi al fine di impedire che da quel varco potessero agire indisturbati gli spacciatori, procurando insicurezza tra i residenti onesti, immigrati e italiani. Più volte il sindaco di Padova ha ripetuto che al completamento dello sgombero delle palazzine seguirà la rimozione della recinzione, perché verranno meno le esigenze per le quali essa è stata realizzata. Successivamente, si potrà passare al risanamento e al recupero urbanistico del quartiere, che prevede, con il coinvolgimento dei proprietari, la diminuzione della cubatura esistente, anche con interventi di demolizione, e soprattutto la realizzazione di alloggi diversificati per tipologia e dimensioni (51 per cento di edilizia residenziale e 49 per cento di uffici e negozi). Il contributo che gli enti locali possono dare per impedire che nelle nostre città si alzino altri muri, molto più problematici, di divisione tra italiani e immigrati, muri che producono esclusione, inquietudine, diffidenza, non può certamente essere separato da una politica nazionale in grado di incoraggiare l'inclusione degli immigrati regolari, la loro integrazione nella vita sociale, economica, politica delle nostre città. Per questo le linee di intervento per l'immigrazione debbono tenere distinte le misure che incoraggiano l'ingresso e la permanenza regolare sul territorio dello Stato, misure praticabili che non possono essere pensate contro l'immigrato che si vuole inserire nella società e che lavora per rendergli ogni giorno la vita difficile, per sospingerlo verso l'irregolarità, da quelle che sanzionano comportamenti illegali, messi in atto dagli immigrati così come da chi favorisce il loro sfruttamento, da chi approfitta dei loro bisogni. Queste linee di intervento - lo ricordava anche il senatore Sacconi - orienteranno il Governo nelle proposte di modifica delle norme attuali, com'è già evidente nei due decreti legislativi all'esame del Parlamento, che, parlando dei ricongiungimenti familiari e dell'abbreviazione del termine per la carta di soggiorno, in linea con le direttive europee, riconoscono all'immigrato alcuni diritti significativi della sua dignità personale e professionale: quello all'unità familiare e quello alla libera circolazione per motivi di lavoro. Due cose mi preme aggiungere rispetto a ciò che ho sentito e che trovo anche

stato realizzato in linea con l'attuale disciplina sull'immigrazione che anche la sua parte politica ha scritto,

al mese di maggio e la cui presentazione ha preso avvio alla data in cui l'allora Governo invitò i datori di lavoro a presentare una documentazione rispetto a

seguire un percorso che, in linea con la legislazione attuale, ha inteso appunto adottare un secondo decreto flussi e non lasciare a terra 350.000 potenziali rapporti di lavoro, che, quando il treno del primo decreto flussi è partito, sono rimasti fermi in un'ipotetica e simbolica stazione. Significa raccogliere le istanze di molti datori di lavoro che sono state espresse anche in occasione della redazione del secondo decreto flussi, in occasione della riunione del gruppo tecnico che ha riferito al comitato ministeriale sulla necessità del decreto stesso; una necessità segnalata, evidenziata, dalle associazioni datoriali così come dalle associazioni sindacali e da quelle di volontariato in occasione di una riunione di quello stesso gruppo. Quindi, a mio avviso, sul piano comunicativo dobbiamo intenderci, perché se dobbiamo chiamare questa «sanatoria», dobbiamo chiamare «sanatoria» anche quella fatta precedentemente dal Governo Berlusconi. Siccome non è così e noi non riteniamo una sanatoria quell'operazione, perché è avvenuta ai sensi di legge, chiediamo allo stesso modo che non si adoperi impropriamente questo termine, che genera confusione nell'opinione pubblica e che quindi è di dubbia correttezza politica e formale, per definire il decreto flussi in corso. Lei diceva, senatore Sacconi, del contratto di lavoro. non ho sentito finora, nelle espressioni del ministro Amato, che si sta pensando a una riforma della legge sull'immigrazione che non leghi la presenza dell'immigrato ad un permesso di soggiorno e ad un rapporto di lavoro. La invito su questo a rileggere insieme le indicazioni che il Ministro ieri ha fornito nel corso dell'audizione in Commissione affari costituzionali qui al Senato. oggi di capire, nell'onestà reciproca, nell'interlocuzione reciproca, come rendere la normativa italiana sempre più in grado di affrontare un fenomeno che è in costante evoluzione, che richiede un dinamismo normativo, che chiede di dirci sinceramente cosa di quelle norme norme non ha funzionato o non sta funzionando e cosa dobbiamo correggere, nell'ottica di un fenomeno che non è emergenziale, ma strutturale, epocale, che ci accompagnerà per tanti anni. Un fenomeno che non è reso soltanto attraverso gli immigrati che sbarcano sulle nostre coste, ma attraverso quella quota consistente di *overstayers* che entrano e restano nel nostro territorio senza un permesso regolare

queste cose ed anche, come sta avvenendo già in Commissione affari costituzionali alla Camera, intorno al disegno di legge sulla cittadinanza. Posso chiederle, Presidente, un minuto, per chiudere su questo punto?

aggiungere all'attuale idea contenuta nelle nostre norme di cittadinanza, un'idea statica, legata prevalentemente allo *ius sanguinis*, un'idea moderna, dinamica, di appartenenza e di condivisione, di chi ha lo *status civitatis*, di un comune tessuto, sociale ed economico. Rispetto a questo, il disegno di legge che il Governo ha presentato ha voluto consegnare un'idea di integrazione, non legata più soltanto ad un fatto temporale, ma legata anche alla verifica, come dice il testo, dell'integrazione sociale e linguistica di chi chiede la cittadinanza. Giudico questa una formula aperta, una formula interessante per un confronto che può

alla differenza, alla distanza che esiste tra le due coalizioni, la maggioranza e l'opposizione, ma si realizzi davvero nella responsabilità, che è comune, di governare un fenomeno e di affrontarlo con serietà nelle sue reali dimensioni

Ringrazio la rappresentante del Governo per la risposta approfondita che ha voluto dare e che, tuttavia, conferma le nostre convinzioni, che mi portano ovviamente a dichiararmi assolutamente insoddisfatto perché, ad ogni livello, la vostra coalizione - in questo caso mi riferisco al Governo del Paese e all**'**amministrazione comunale di Padova - offre purtroppo il il contesto più idoneo per il manifestarsi di quelle patologie che rischiano di diffondersi e di produrre diffusamente condizioni di «disintegrazione». Mi riferisco, nel caso dell'amministrazione comunale di Padova, ad un complesso di azioni alle quali quell'amministrazione si è dedicata più intensamente che non al risanamento e alla bonifica di via Anelli**:** all'idea di una moschea nella città, all'idea di ammettere in Consiglio comunale il Presidente della Consulta degli immigrati, all'idea di consegnare il voto agli immigrati per le elezioni di quartiere. Nel caso stesso delle azioni di bonifica, è in corso un contenzioso tra l'amministrazione comunale e l'ATER, citato anche dal Sottosegretario, a proposito della competenza in ordine al ricollocamento degli inquilini, nascondendo questo conflitto, da un lato, una volontà di esercizio del potere connesso per ragioni evidentemente di cattura del consenso, e dall'altro, forse, anche un non sufficiente rigore nel distinguere soggetti regolari da soggetti irregolari. Insisto: non dimentichiamo che nella stessa città di Padova coloro che nei giorni scorsi sono stati protagonisti di scontri sono parte esplicita, dichiarata della coalizione che governa quella città e hanno persone che ritengono di rappresentarli probabilmente anche all'interno della stessa Giunta comunale.

un atto che interviene sostanzialmente dopo la programmazione dei flussi, a seguito della presentazione delle domande, e che porta le quote da 99.500 unità del 2005 a ben 520.000? Che cos'è questa, se non un'operazione a piè di lista? Vogliamo chiamarla regolarizzazione, vi è più dolce la definizione? Essa è comunque un'operazione a piè di lista, che significa rinuncia a selezionare i flussi in ragione della sostenibilità dei rapporti di lavoro. Questa è una ragione non secondaria che, per esempio, portò il nostro Governo ad accogliere *in* *toto* le domande stimate per gli assistenti familiari, ma non *in* *toto* le domande relative, ad esempio, ad operai manifatturieri, non ritenendo quella professionalità tale da essere sostenibile nel tempo. Ne sappiamo qualcosa io e il senatore Stiffoni per quanto riguarda una nota azienda che ha rimesso recentemente nel mercato del lavoro molti cittadini immigrati per i processi di riconversione e ristrutturazione che sono in corso. Per quanto riguarda - e ho finito alla cittadinanza, vorrei ricordare che il giudizio pesantemente negativo che noi diamo su di esso è fondato proprio sul fatto che esso si collega a flussi subiti e che, non solo per il passato ma anche per il futuro, c'è un combinato disposto tra flussi subiti e riconoscimento, così agevolato, dei diritti di cittadinanza. Tali diritti sono - ricordiamolo - diritti di sovranità che richiedono condizioni molto più accorte per essere concessi, anche alla luce dei fenomeni di pericolo per la stessa sicurezza nazionale.

sono gli ambiti in cui semmai si dovrebbe intervenire per migliorare e ottimizzare la spesa pubblica, in sostanza per risparmiare sulla spesa e sui sacrifici che chiediamo ai contribuenti. L'interpellanza però tocca un ambito

così smisurati; è difficile capire come possono essere utilizzati. Presuppongo ci sia un errore nell'uno o forse nell'altro dato. Se ci è consentito un vezzo, abbiamo provato a paragonare il Quirinale con la Casa Bianca; Bianca; presso il Quirinale sembra siano in dotazione circa 40 auto di servizio.

non sembra siano fornite al titolare esclusivamente per funzioni di servizio, ma sembrano assegnate addirittura *ad personam*, con un uso *ad libitum*, discrezionalissimo, sia per lavoro, sia per diporto, sia per altri utilizzi. Quello che l'interpellante esprime è che, dopo averlo sentito nelle dichiarazioni programmatiche di questo Governo, sarebbe anche ora di vedere qualcosa muoversi in questo senso e cioè un ridimensionamento dei mezzi Stato a disposizione, per esempio, di soggetti decaduti dalle cariche e non più necessitanti pertanto di visibilità, di strutture, di mezzi di dotazione della pubblica amministrazione. Come bisognerebbe magari anche ripensare lo stesso impiego dei famosi funzionari di alto rango. Premesso quanto detto, l'interpellante rivolge alcune domande precise al rappresentante del Governo, proprio sulla base delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio. Visto che Prodi ha ritenuto di far presente a tutti i Ministri di ridurre drasticamente queste spese, si chiede in quale misura a questo punto - il rappresentante del Governo ce lo potrà dire - si riterrà di operare riduzioni

Altra questione su cui ci sta a cuore avere risposte è per quanto tempo, secondo voi, un soggetto che non ricopre più cariche pubbliche dovrebbe beneficiare degli attuali servizi messi a disposizione.

prestazione da parte dello Stato ai soggetti non più in carica. considerando - richiamiamoci alle dichiarazioni del Ministro dell'economia e delle finanze - che il tutto è incompatibile, del resto, con lo stato delle finanze di questo Paese.

citare un caso su tutti, proprio perché emblematico: l'onorevole Pivetti, cessata dalla carica di Presidente della Camera all'età di circa trenta'anni, godrà di un trattamento privilegiato

ha colto e ha ricordato un aspetto fortemente presente nelle premesse e nell'azione di questo Governo, che riguarda essenzialmente il tema della complessiva riduzione dei costi della politica e di una incisiva lotta agli sprechi, tema che, come è detto nell'interpellanza, riguarda, anche se non solo, la questione delle cosiddette auto blu. A questo obiettivo di una riduzione si può pervenire anche a legislazione invariata, a legislazione invariata, attraverso una capillare revisione delle singole situazioni per verificarne l'attualità e la congruità rispetto alle disposizioni vigenti e più in particolare la permanenza dei presupposti oggettivi e soggettivi che danno luogo all'assegnazione delle autovetture di servizio. Per quanto riguarda lo Stato, una strategia di contenimento in tal senso è già in atto ed è intendimento del Governo implementarla ulteriormente, anche in coerenza con quell'indirizzo di riduzione dei costi più volte annunciato dal Presidente del Consiglio e richiamato dall'interpellante. L'auspicio è che alla stessa finalità - in questo senso raccolgo la parte che ci compete, ma è evidente che le cifre comprendono altri soggetti, altri livelli, altre istituzioni altri livelli, altre istituzioni - possano ispirarsi anche le iniziative che le altre dimensioni territoriali di Governo potranno assumere nel rispetto della loro autonomia organizzativa. Com'è noto, nel sistema attuale l'assegnazione di autovetture di servizio ai titolari di determinati uffici pubblici avviene sulla base dei criteri stabiliti da specifiche previsioni normative, che stabiliscono, tra l'altro, le categorie dei possibili beneficiari ed i limiti di durata del beneficio. Ricordo, in particolare, le disposizioni dell'articolo 2, comma 118 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, Consiglio dei ministri. 30 ottobre 2001, relativamente alle «assegnazioni in uso esclusivo delle autovetture di servizio delle Amministrazioni civili dello Stato» e quelle della direttiva del 30 ottobre 2001 del Ministro per la funzione pubblica, specificamente concernente «modi di utilizzo delle autovetture di servizio delle Amministrazioni civili dello Stato e degli enti pubblici non economici». Il vincolo che lega l'assegnazione del veicolo all'assolvimento di un determinato incarico comporta che la cessazione di quest'ultimo determini la decadenza della stessa assegnazione - questo è un punto di risposta preciso ad un suo quesito - come avvenuto, ad esempio, per i Sottosegretari del Ministero dell'interno del precedente Governo non destinatari di misure di protezione. Diversa è la situazione per quelle personalità le quali, pur non ricoprendo più incarichi attivi di Governo, sono tuttora sottoposte a scorta o tutela per esplicita previsione di legge, ovvero per la permanenza di un'elevata esposizione al rischio. In questo caso, la cosiddetta auto blu non è evidentemente un'autovettura di servizio, bensì un veicolo assegnato per l'attuazione del dispositivo di protezione ravvicinata. Nel caso del Ministero dell'interno, l'autoparco del Dipartimento di pubblica sicurezza ha in dotazione 1.420 veicoli, ivi comprese le autovetture blindate, molti dei quali, oltre che nell'ambito dei dispositivi di protezione delle persone sottoposte a pericoli per la propria sicurezza personale, sono assegnati alle varie direzioni centrali e agli uffici periferici per l'assolvimento di compiti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, ovvero per altre esigenze istituzionali o di servizio. Di queste, circa 400 sono utilizzate per l'esecuzione di misure di protezione personale. A questo proposito, ricordo che il relativo sistema, che è stato completamente riorganizzato secondo le disposizioni del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 2002, n. 133, stabilisce in modo rigoroso i presupposti ed il procedimento per l'adozione di dispositivi di tutela, graduandone l'intensità in relazione all'effettivo grado di rischio riscontrabile in ciascuna situazione. Pertanto, a parte, come detto, un ristrettissimo numero di personalità istituzionali individuate in ragione della carica rivestita e del rischio insito nell'alto livello di esposizione, per le quali la protezione personale è stabilita direttamente dalle disposizioni vigenti, per tutti gli altri soggetti l'adozione delle misure tutorie è subordinata ad una approfondita valutazione di carattere tecnico, tesa a verificare, caso per caso, l'effettiva sussistenza di un pericolo o di una minaccia per l'interessato ed i suoi familiari, secondo i criteri stabiliti dalle stesse norme. In quanto strettamente correlati all'attualità della situazione di pericolo, i dispositivi di protezione, una volta decisi, sono soggetti a periodica revisione e ad un monitoraggio costante. Segnalo, infine, che il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, relativamente alla gestione dei veicoli, ha realizzato, nel primo semestre dell'anno in corso, un contenimento della spesa superiore al 10

per fortuna, il campo nomadi a Treviso non c'è più, e lei lo sa benissimo. Erano anni che noi, come amministrazione comunale, tentavamo di porre rimedio a questa disastrosa situazione. Ma il punto della mia interrogazione non è tanto questo, anche perché l'ho presentata immediatamente a seguito del mancato sgombero di quel campo nomadi. Tutto era stato predisposto da mesi, per non dire da anni. Vi è un'informativa del 10 luglio del questore di Treviso - che lei conosce benissimo quale ribadisce appunto che mercoledì 12 luglio, dalle ore 7 del mattino, si sarebbe provveduto allo sgombero del campo nomadi, quando tutto - lei sa benissimo - era stato già predisposto. Addirittura, alcuni nuclei familiari, con o senza le loro *roulotte*, se ne erano già andati. Già dal mattino, ancora prima delle 7, alcuni avevano cominciato a fare i propri bagagli per andarsene. Tutto era stato predisposto dall'amministrazione comunale al punto che si era già preso contatto con una serie di alberghi di Treviso per ospitare queste famiglie nomadi. Questo, signor Presidente, per creare l'emergenza abitativa: abitativa: per bypassare certe disposizioni contenute nella disciplina dell'assegnazione degli alloggi delle case popolari, bisognava provvedere allo sgombero e creare l'emergenza abitativa.

alle 100-150.000 lire del vecchio conio; non era una sistemazione da disprezzare. Tutto era stato predisposto, tutto era a conoscenza sia del prefetto che del questore:

una decina dei quali già avevano abbandonato il campo. Vorrei sottolineare, signor Presidente, come sa benissimo il rappresentante del Governo, che non tutti questi nuclei familiari avevano la residenza a Treviso. Alcuni l'avevano in altri posti.

dopo una settimana è cominciata e si è conclusa positivamente nel giro di una quindicina o ventina di giorni. Ma cosa è successo quel giorno? Improvvisamente è arrivato il questore questore nella sede del campo nomadi verso le ore 13 e, con motivazioni assurde, completamente in contrasto con quello che aveva scritto lui stesso il 10 luglio, cioè due giorni prima, bloccava

che si creasse quell'emergenza abitativa e quella catena che avrebbe portato all'assegnazione, da lì a pochissimi giorni, degli alloggi. Già tutte le abitazioni erano state individuate e segnalate,

sapere se sia stata un'iniziativa deprecabile da parte del questore di Treviso, in unione con il prefetto, oppure se certe disposizioni e suggerimenti siano pervenuti a Treviso direttamente dal Ministero.

questa data sono state, infatti, trasferite dodici famiglie di nomadi scinti in alloggi messi a disposizione dell'amministrazione comunale. si era reso necessario per motivi di ordine pubblico, in quanto nella data precedentemente fissata, al momento fissata, al momento di procedere allo sgombero, era emersa una forte resistenza di alcuni dei nuclei familiari interessati che non intendevano accettare la nuova sistemazione alloggiativa.

ricollocazione delle famiglie in alloggi di edilizia popolare, proprio alla vigilia delle operazioni la stessa amministrazione aveva indicato, come unica soluzione immediatamente praticabile nell'ottica della dichiarazione di emergenza abitativa, quella di una provvisoria sistemazione in albergo; di questo però gli interessati

Infatti, tale circostanza, insieme alle insufficienti informazioni circa la garanzia di una successiva e rapida assegnazione degli alloggi, ha alimentato preoccupazioni e opposizioni allo sgombero tra le famiglie interessate dal provvedimento in questione. tener conto - questo lo ricorderà, senatore Stiffoni - che a Treviso, già in passato, analoghe operazioni di sgombero avevano determinato problemi di ordine pubblico, ad esempio nel 2003, quando gruppi di nomadi e stranieri occuparono per protesta il sagrato del duomo cittadino. Si è pertanto ritenuto più opportuno riprogrammare a breve termine lo sgombero non appena si fossero realizzate tutte le condizioni perché esso potesse svolgersi serenamente,

erano perfettamente a conoscenza e tutte avevano accettato. Non è assolutamente vero che ci siano stati dei moti particolari per contrastare

l'interno*. Rispondendo all'interrogazione del senatore Iovene sulla situazione della sicurezza pubblica in Calabria, in particolare nella città di Lamezia Terme, voglio intanto ribadire il sostegno del Governo a tutti coloro che in Calabria lavorano e rischiano la vita per difendere la legalità, la democrazia e il diritto a vivere liberi dalla paura e dal bisogno. La questione calabrese è seguita con la massima attenzione dal Ministero dell'interno ed è stata oggetto di numerosi incontri con parlamentari di tutte le parti politiche, con amministratori locali, con qualificati esponenti del mondo economico e del lavoro, al fine di trovare ed attuare una strategia comune d'intervento. Negli ultimi anni, e in particolare dal luglio 2004, di fronte all'aggravarsi degli atti intimidatori nei confronti di amministratori pubblici e di imprenditori calabresi, che mettevano in evidenza un incremento dell'invasività della 'ndrangheta nel tessuto socio-economico, è stata avviata un'approfondita analisi sulle cinque province calabresi al fine di implementare l'azione di prevenzione e di contrasto nei confronti della criminalità organizzata calabrese. Tale attività si è conclusa con la Conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza del 30 luglio 2004 a Catanzaro, dove è stato concordato un programma articolato in tre fasi. La prima fase ha previsto un rafforzamento dell'attività di controllo del territorio e di quella investigativa; la seconda, un collegamento più stretto con l'autorità giudiziaria finalizzato ad accelerare la fase esecutiva delle attività investigative in atto; la terza, un'elevazione degli *standard* di sicurezza con interventi tecnologici. Come sappiamo, dopo l'omicidio del vice presidente della Regione Francesco Fortugno, avvenuto il 16 ottobre 2005, è stato ulteriormente sviluppato il programma straordinario di intervento nella Regione Calabria, che prevede varie linee d'azione, tra cui l'intensificazione dei dispositivi di sorveglianza e di controllo del territorio calabrese, il rafforzamento di tutte le attività informative ed investigative, con l'applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali, il controllo di tutte le operazioni antidroga e la tutela degli amministratori locali. Tale strategia sta producendo risultati significativi, grazie all'impegno congiunto della magistratura e delle forze di polizia. In particolare, si è giunti all'arresto degli esecutori materiali e, con l'operazione del 21 giugno scorso, dei presunti mandanti dell'omicidio Fortugno. Nell'arco di circa due anni, l'azione di contrasto ha consentito i seguenti risultati: l'arresto di oltre 6.000 persone, tra cui 50 latitanti, di cui 5 inseriti nel «programma speciale di ricerca dei 30 latitanti più pericolosi» e sette nell'«opuscolo dei 500»; la disarticolazione di 30 associazioni di tipo mafioso e 19 sodalizi criminali dediti al traffico di sostanze stupefacenti; la repressione di gravissimi episodi illeciti nel settore dei finanziamenti pubblici comunitari, nazionali e regionali; il sequestro, in materia di contrasto ai reati inerenti agli stupefacenti, di 340.000 piante di canapa indiana; la proposta di 467 misure di prevenzione personali e di 40 patrimoniali; l'applicazione dell'articolo 12-*sexies* della legge n. 356 del 1992, che ha sottratto alla criminalità organizzata calabrese beni ed immobili per oltre otto milioni di euro. Le iniziative di contrasto avviate hanno prodotto risultati importanti anche nel territorio lametino. Nel mese scorso, due distinte operazioni di polizia giudiziaria hanno rapidamente consentito l'identificazione ed il fermo, quali indiziati di delitto, di tre elementi di una famiglia mafiosa locale, ritenuti responsabili di due omicidi consumati il 28 luglio ed il 4 agosto scorsi. Le stesse strutture investigative, nel mese di giugno, avevano identificato e sottoposto a fermo, quale indiziato di delitto, un altro pregiudicato locale affiliato ad una cosca del catanzarese, per un tentato omicidio perpetrato nelle campagne di Pianopoli. I predetti fermi sono stati tutti convalidati dall'autorità giudiziaria. Altri risultati di rilievo sono stati raggiunti sul fronte del contrasto al fenomeno estorsivo in danno di imprenditori ed altri operatori economici della zona. In particolare, sono stati tratti in arresto, per estorsione aggravata, quattro affiliati ad una cosca lametina e denunciati a piede libero, per lo stesso titolo di reato, altri elementi della stessa consorteria criminale. Si tratta, come detto, di risultati significativi che tuttavia non esauriscono, evidentemente, l'impegno degli apparati dello Stato per combattere la criminalità organizzata in Calabria, impegno che, al contrario, continuerà a dispiegarsi con la massima dedizione e determinazione. Per dare il senso dell'ampiezza degli interventi da realizzare, ricordo che nell'ambito del «programma Calabria» sono stati presentati progetti per la realizzazione di sistemi per la videosorveglianza di centri urbani, arterie di collegamento di interesse strategico e insediamenti produttivi; in tutte le Province sono stati istituiti appositi tavoli permanenti o, comunque, si sono svolti incontri con i rappresentanti istituzionali e del tessuto produttivo, in tema di estorsioni e di atti intimidatori nei confronti di pubblici amministratori ed imprenditori. Gli interventi dello Stato, volti a sostenere lo sviluppo economico dell'area, sono affiancati da un rafforzamento delle misure di tutela della sicurezza pubblica. In tale ottica, è stato attivato il Patto territoriale del lametino come strumento di concertazione tra le diverse forze sociali interessate, al quale è annesso un Protocollo di legalità che prevede, altresì, la costituzione di un Osservatorio relativo agli appalti sui lavori pubblici. Inoltre, a seguito dell'Accordo di programma quadro a suo tempo sottoscritto nell'ambito del Programma operativo nazionale «Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia», il 30 maggio scorso è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa tra il presidente della Regione Calabria, il prefetto di Reggio Calabria ed il prefetto di Catanzaro con lo scopo di verificare l'attuazione delle forme di collaborazione avviate tra Stato e Regione per rafforzare l'azione di contrasto all'illegalità. In questo contesto, il coordinamento delle azioni e degli interventi rappresenta un elemento fondamentale della strategia condotta e ha trovato una sua concreta traduzione in vari momenti di confronto, di raccordo e di scambio conoscitivo. In particolare, il 16 giugno scorso, presieduta dal direttore centrale della Polizia criminale, si è svolta a Roma una riunione tecnica sugli episodi delittuosi che hanno investito la Calabria ed il lametino in particolare, alla quale hanno partecipato il direttore della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, il direttore della Direzione investigativa antimafia ed il direttore della Direzione centrale per i servizi antidroga, nonché qualificate rappresentanze dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Successivamente, il 19 giugno, il vice ministro dell'interno, onorevole Minniti, ha presieduto a Reggio Calabria i lavori della Conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza, dedicata, in particolare, agli aspetti attuativi del piano di interventi straordinari in corso. Durante l'incontro c'è stata una larghissima convergenza su alcune questioni fondamentali ed, in primo luogo, sul tema della sicurezza in Calabria, che non è un problema solo dei calabresi, ma costituisce una variante del tema della sicurezza dell'intero Paese. Si è convenuto, inoltre, che la lotta alla criminalità organizzata costituisce una priorità assoluta delle politiche di Governo nazionale e come tale richiede programmi e strategie in grado di attivare una concorde sinergia fra politica, magistratura e amministrazione. La riunione ha consentito di operare una disamina delle principali attività e degli impegni già in atto, concernenti tutte le componenti interessate, e di delineare una mirata azione di risposta da parte dell'apparato di sicurezza statale con una pianificazione di una rinnovata strategia investigativa, volta a perfezionare le misure in corso attraverso un'ulteriore valorizzazione di tutte le diverse professionalità dispiegate dai vari organismi di polizia, in un quadro di funzionale condivisione anche con le competenti autorità giudiziarie. Un successivo incontro, svoltosi il 20 giugno presso la sede del centro DIA di Catanzaro, ha permesso di focalizzare in modo specifico il tema del coordinamento delle attività d'indagine relative agli ultimi omicidi verificatisi nel comprensorio lametino. All'incontro, a cui hanno preso parte il procuratore della Repubblica di Catanzaro e magistrati della Direzione distrettuale antimafia, sono intervenuti i responsabili delle articolazioni operative periferiche delle forze di polizia, dei servizi interprovinciali e della DIA. In quell'occasione, esaminate le risultanze, sono stati condivisi i criteri da seguire per l'ulteriore sviluppo dell'attività investigativa, stabilendo mirate deleghe d'indagini ad appositi gruppi di lavoro distinti per forza di polizia, assegnando a ciascun organo l'approfondimento degli accertamenti nei confronti degli ambienti legati a specifiche cosche criminali e prevedendo un costante interscambio informativo, per costituire una piattaforma di conoscenze comuni. Per quanto concerne gli specifici aspetti evidenziati dal senatore Iovene, assicuro, quindi, che per gli omicidi del 31 marzo e 12 maggio scorso perpetrati a Lamezia e Feroleto, così come per gli atti intimidatori consumati ai danni di esercenti, imprenditori e pubblici amministratori, sono in corso attivissime indagini condotte, d'intesa con l'autorità giudiziaria, da investigatori della Sezione criminalità organizzata della Squadra mobile di Catanzaro e del commissariato di Lamezia Terme. Quanto all'attività di prevenzione anticrimine e controllo del territorio, essa è stata potenziata con l'impiego complessivo, dal 1° gennaio al 12 settembre del corrente anno, di 593 equipaggi del Reparto prevenzione crimine Calabria e con lo svolgimento di numerose perquisizioni domiciliari e controlli straordinari a carico di persone sottoposte a misure limitative della libertà personale. E' stato, altresì, intensificato il numero di pattuglie da parte del Comando regionale carabinieri Calabria e di altre compagnie del Comando provinciale dei carabinieri, con la conseguente presenza contemporanea sul territorio di Lamezia Terme di cinque-sei pattuglie durante l'arco delle ventiquattr'ore a fronte delle due-tre pattuglie impegnate in precedenza. Si tratta di un impegno che denota la particolare attenzione rivolta ad un territorio con un indice di delittuosità superiore a quello nazionale (4.910 delitti ogni 100.000 abitanti, contro 4.052). Ricordo, infine, che il numero di operatori delle forze di polizia presenti nel Comune di Lamezia Terme risulta pari a 504 unità, delle quali 243 per la Polizia di Stato, 95 per l'Arma dei carabinieri e 166 per la Guardia di finanza. Il rapporto tra popolazione e forze di polizia risulta risulta quindi di un operatore ogni 140 abitanti, più favorevole di quello relativo alla Regione Calabria (un operatore ogni 175 abitanti) e a quello relativo all'intero territorio nazionale (un operatore ogni 256). Tale dato, unitamente agli importanti risultati ottenuti sul piano informativo ed investigativo, ci porta a ritenere adeguata l'attuale consistenza dei presìdi delle forze di polizia presenti a Lamezia Terme. Nondimeno, in considerazione dell'andamento della criminalità nella zona, le istanze per un loro ulteriore potenziamento vengono tenute presenti per un'eventuale e successiva rivalutazione che tenga conto delle esigenze complessive della sicurezza pubblica nell'intero territorio calabrese.

Prendo atto, quindi, positivamente del programma di azione e contrasto alla criminalità organizzata che il Governo intende seguire per quanto riguarda la Calabria. Voglio però sottolineare che il Comune di Lamezia Terme, ormai la terza città della Calabria, è stato sciolto per infiltrazioni mafiose due volte in dieci anni, che dopo le ultime elezioni amministrative il primo biglietto da visita che la criminalità organizzata ha presentato al nuovo sindaco è stato l'incendio del portone del municipio (da allora il sindaco è costretto a vivere sotto tutela) che, nonostante i risultati apprezzabili dal punto di vista delle indagini e delle attività giudiziaria che sono stati qui ricordati, purtroppo i fatti delittuosi continuano verificarsi e sono assai gravi: non solo omicidi, ma anche atti estorsivi e altri episodi di criminalità organizzata. Quindi, più che un problema di quantità c'è un problema di qualità delle indagini e anche la necessità di un maggiore coordinamento dell'azione delle delle forze di polizia e di queste con l'autorità giudiziaria. Vi è poi la necessità di un ulteriore cambio di passo, di un'accelerazione. di un'accelerazione. Lamezia Terme, come Locri, è un'area particolarmente calda della Calabria e necessita di una particolare attenzione, ed è questo l'intento che voleva raggiungere l'interrogazione, che qui confermo e sollecito.

Si tratta però di dare risposte anche con fatti simbolici: la caserma dei Carabinieri è praticamente chiusa perché pericolante da

nella Provincia di Caserta è significativa la presenza di organizzazioni criminali di nazionalità extracomunitaria ormai radicate sul territorio, che si sono aggiunte ai sodalizi criminali locali, fra i quali quello egemone dei Bidognetti. Al momento, è in corso un processo che si può definire di assimilazione poiché la delinquenza extracomunitaria delle varie etnie mantiene collegamenti con la criminalità organizzata dei Paesi di origine, operando parallelamente ai sodalizi locali, che delimitano, e in qualche modo garantiscono, l'operato della criminalità extracomunitaria. In particolare, nella zona di Castel Volturno, la situazione è cominciata a degenerare a partire dal 1980 quando, in seguito al sisma che colpì gravemente varie zone della regione Campania, furono requisiti numerosi edifici ubicati lungo il litorale per destinarli a coloro che erano stati gravemente danneggiati dall'evento. La condizione di grave degrado che ne seguì ha favorito, grazie ai bassi livelli dei canoni di locazione degli edifici ridotti in pessimo stato dagli occupanti, l'insediamento di numerosi cittadini extracomunitari (dei quali, allo stato attuale, 1.500 regolari ed un numero di irregolari quantificabile in oltre 1.500 unità) prevalentemente di origine nigeriana e albanese. La delinquenza nigeriana è particolarmente attiva, oltre che nel settore del narcotraffico, nel controllo della prostituzione di giovani donne connazionali. Anche la malavita organizzata albanese ha rivolto la propria attenzione al mercato della droga, al traffico degli esseri umani e allo sfruttamento della prostituzione. Sulla base dei dati disponibili alla data del 1° agosto scorso, sul territorio della Provincia di Caserta risultano dispiegati complessivamente 2.520 operatori di pubblica sicurezza rispetto ad una forza organica di 2.536 unità, con una differenza d'insieme tra gli organici e gli effettivi di 16 unità. L'ordinario dispositivo di controllo del territorio si avvale, peraltro, dell'ausilio costante del Reparto prevenzione crimine Campania della Polizia di Stato che, dal 1° gennaio al 30 giugno del corrente anno, ha impiegato 481 equipaggi. Nell'ambito della pianificazione delle risorse disponibili per l'anno 2005, è stata già disposta l'assegnazione alla questura di Caserta di 10 appartenenti alla Polizia di Stato, mentre, con riferimento alla programmazione di quelle disponibili per il corrente anno, l'esigenza della Provincia verrà attentamente valutata compatibilmente con le priorità delle altre realtà territoriali. Inoltre, per effetto dei piani per i rinforzi estivi per il 2006, che rappresentano lo sforzo più elevato espresso dalle forze di polizia per soddisfare - a livello nazionale - le esigenze di sicurezza delle località maggiormente interessate dall'afflusso turistico, sono stati assegnati 30 militari dell'Arma dei carabinieri, in aggiunta al personale in forza ai presìdi territoriali distribuiti nella predetta Provincia. Nel territorio del Comune di Castel Volturno operano un commissariato di pubblica sicurezza ed una stazione dell'Arma dei carabinieri. Nel primo prestano servizio 51 appartenenti ai ruoli operativi della Polizia di Stato rispetto alla previsione organica di 47 unità, cui devono aggiungersi due appartenenti all'amministrazione civile dell'interno che, nei settori di supporto logistico e burocratico, contribuiscono alla funzionalità delle strutture. La stazione dei Carabinieri è, invece, dotata di una forza effettiva di 19 militari, superiore di un'unità rispetto alla previsione organica, e si avvale, in occasione di specifiche azioni di repressione della criminalità, di militari delle compagnie di Mondragone (CE) e di Casal di Principe

Di uguale rilievo sono stati i risultati raggiunti dalla Polizia di Stato che, nel corso del 2006, ha condotto a termine importanti operazioni nei confronti di esponenti malavitosi del *clan* egemone dei Bidognetti, con l'arresto di due elementi di spicco e di altri 35 appartenenti al sodalizio criminoso, nonché con la cattura di un noto latitante. Tali operazioni, frutto di una costante attività investigativa, costituiscono il segno tangibile dell'efficacia dell'azione di contrasto svolta dalle Forze di polizia, che ha contribuito a stemperare l'aggressività dei sodalizi criminali. Oltre all'attività di repressione, sono stati intensificati da tempo i servizi di controllo straordinario del territorio anche in orario serale, finalizzati al contrasto di gravi reati, tra i quali la tratta degli esseri umani volta allo sfruttamento della prostituzione di cittadine extracomunitarie e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Per quanto riguarda l'utilizzo di manodopera straniera in agricoltura, risulta effettivamente che nel territorio di Castel Volturno è frequente il ricorso a braccianti di nazionalità prevalentemente indiana e nordafricana per il lavoro nei campi. Il tema del contrasto del lavoro nero degli immigrati è ben presente all'attenzione del Governo, tant'è che il 5 settembre scorso il Ministro dell'interno ha istituito una commissione, presieduta dal capo della Criminalpol, alla quale ha affidato l'incarico di verificare in tempi brevi le situazioni di illegalità connesse allo sfruttamento dei lavoratori extracomunitari. La commissione concluderà i suoi lavori agli inizi del mese di ottobre e il Ministro dell'interno ha già assunto l'impegno di riferire subito dopo in Parlamento per illustrare le conclusioni raggiunte. Nello stesso tempo, sempre su indicazione del Ministro, è stata posta allo studio una modifica dell'articolo 18 del Testo unico sull'immigrazione, che prevede una speciale tutela per gli stranieri clandestini sfruttati da parte di organizzazioni criminali sotto inchiesta per reati di particolare gravità. In sede locale, per seguire attentamente l'andamento del fenomeno, sono stati costituiti gruppi ispettivi misti, composti da operatori delle Forze dell'ordine e da rappresentanti dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Caserta, dell'INPS e dell'INAIL, con il compito di svolgere operazioni di controllo nelle aziende agricole verificare eventuali irregolarità sull'assunzione dei lavoratori e l'esistenza di situazioni di sfruttamento. Il problema ha formato anche oggetto di indagine della locale Squadra mobile. Gli accertamenti esperiti, pur non facendo emergere veri e propri fenomeni di caporalato, hanno invece consentito di deferire all'autorità giudiziaria, negli anni 2005-2006, circa 90 persone, di cui 10 italiane, ritenute responsabili di concorso in false attestazioni e favoreggiamento della permanenza sul territorio nazionale di cittadini stranieri irregolari. Proprio nella settimana scorsa, nella zona di Mondragone, confinante con quella di Castel Volturno, sono state denunciate in stato di libertà all'autorità giudiziaria, per i fatti indicati, quattro persone di cittadinanza italiana. Grazie ai finanziamenti del Programma operativo nazionale «Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia», sono stati realizzati, anche per la città e la provincia di Caserta, importanti interventi tecnologici per la razionalizzazione del dispositivo di controllo del territorio. Sono stati portati a termine il progetto «Sale Operative» della Polizia di Stato e dei Carabinieri, cui si andranno ad aggiungere quelle della Guardia di finanza, per migliorare il sistema di prevenzione e per l'impiego di pattuglie per il controllo del territorio; il progetto «SIDAF - Sistema Informativo per il Controllo delle Frontiere», per l'acquisizione di apparecchiature per il controllo dei passaporti e l'identificazione delle persone in entrata e uscita dal territorio nazionale ed europeo; il progetto «Potenziamento Gabinetti provinciali» della Polizia scientifica, al fine di migliorare l'efficacia dell'azione investigativa della Polizia di Stato attraverso l'acquisizione di nuove strumentazioni; il progetto «AFIS - Uffici Periferici», per l'adeguamento tecnologico dei collegamenti al Casellario centrale d'identità. Sono state acquisite tecnologie di nuova generazione per il controllo delle reti e degli assi viari, del territorio e delle frontiere aeree, marittime e terrestri, nonché per il contrasto all'immigrazione clandestina e la tutela ambientale. Per l'ottimale impiego dei predetti apparati, sono stati finanziati corsi per la formazione avanzata del personale delle forze dell'ordine sull'utilizzo delle tecnologie informatiche nel settore delle indagini informatiche e delle reti telematiche.

atto, infatti, al Governo di cogliere la pericolosità della complessiva situazione che si è determinata in provincia di Caserta, in particolare nell'area di Castel Volturno, che vede la confluenza di presenze criminali locali e straniere, quest'ultime facenti parte dell'immigrazione che sta prendendo piede nelle attività criminali della zona. Sicuramente è un punto sul quale sul quale è assai importante che ci sia una presa di coscienza, anche se poi dai numeri che il Governo

pensare che con questo tipo di forze si riesca a contrastare una presenza criminale che sta diventando veramente importante qualche dubbio può generarsi.